L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

una richiesta popolare, promossa dall'Assessorato alle politiche sociali e pari opportunità della Provincia di Treviso e sottoscritta da oltre duemila uomini e donne dello stesso territorio in soli due giorni, affinché l'attuale Governo, del quale

al fine di continuare l'azione di contrasto e prevenzione al fenomeno della violenza sulle donne e, al contempo, si impegni nel presentare un disegno di legge che garantisca alle donne, sul piano dei diritti civili Il divario che separa l'Italia dagli altri Paesi dell'Unione europea mostra che, in ambito occupazionale, è tale la disparità di trattamento tra uomini e donne da meritare

a criteri di necessità ed urgenza e, in quanto tale, non ha i presupposti per affrontare un fenomeno sociale e culturale così complesso e di così ampia portata. L'iniziativa che sottopongo alla Presidenza del Senato è volta a sostenere l'impegno già dimostrato dal Governo in tal senso, sollecitando lo stesso a proseguire in questa direzione con un'azione ancora più incisiva,

Senatore Stiffoni, certamente la sua richiesta sarà trasmessa al Presidente del Senato.

con la grande maggioranza dei suoi membri, che fa parte tra l'altro del più vasto intergruppo parlamentare a sostegno del Tibet, una mozione con cui si chiede al Governo italiano di farsi portatore di alcune richieste del Dalai Lama e del Governo tibetano in esilio in seno alle Nazioni Unite: *in primis*, l'accesso a osservatori internazionali indipendenti per verificare ciò che accade e, in secondo luogo, rendere noto al mondo cosa in effetti il Dalai Lama chiede a Pechino, cioè non l'indipendenza, ma un'ampia autonomia politica. In Senato non siamo riusciti a portare avanti la stessa iniziativa, a causa di altri tipi di urgenze ed emergenze che hanno caratterizzato i nostri lavori. Tuttavia, dato che quest'anno ricorre anche il ventesimo anniversario di un'altra

Malpensa e Fiumicino. In tal modo, sarà possibile scegliere una compagnia che funziona, rispetto all'altra che oggettivamente non funziona. Questo, al di là di garantire una funzionalità - mi scusi il bisticcio - del Senato (se oggi si fosse iniziato alle ore

questione molto delicata che attiene proprio all'ordine dei lavori, ovvero ad un'interrogazione parlamentare che gli Uffici hanno respinto, affermando che alcune autorità

L'interrogazione, che è stata respinta perché ci sarebbe una prassi in tal senso, riguarda il bando di gara, di durata triennale, approntato dalla Banca d'Italia per la fornitura di servizi di ristorazione al costo modico di 24.500.000 euro, prorogabile per altri due anni, per un totale di 41.500.000 euro. All'interno del bando e dei relativi allegati (di ben 450 pagine) sono previsti nel dettaglio, in controtendenza con la profonda crisi che sta investendo l'intero Paese, vari tipi di pregiatissimi menu, divisi per importanza, stagione, settimana e festività, compresi il servizio camerieri e *maître* di coordinamento, il servizio bar e caffetteria, con la precisazione del marchio desiderato e i vari tipi di bevande richieste; il tutto ad altissimo standard, per l'ammontare di 34.500 euro al giorno.

la propria cultura, le proprie tradizioni, le proprie forme di vita e di sviluppo. È giusto altresì sottolineare che quanti si battono a questo fine richiedono, a partire dal Dalai Lama,

Garavaglia e la senatrice Biondelli hanno invece denunciato il forte disagio che riguarda tutti i cittadini rispetto al funzionamento di Alitalia. Anche questo può essere portato, come tema specifico di indirizzo politico, al confronto della Commissione competente e dell'Assemblea con gli strumenti di sindacato ispettivo. Il senatore Garavaglia ha posto anche un'altra questione concernente

il motivo per cui gli Uffici hanno sollevato l'eccezionerispetto alla sua interrogazione è il

definitivamente l'intrusione dei vari partiti che legittimano un voto non lecito, perché espresso da persone che mettono le mani su più

aveva escluso il ricorso al voto attraverso le impronte digitali. Le ricordo che in quest'Aula è stata introdotta, a differenza delle precedenti legislature, la postazione fissa per i senatori.

all'emanazione di un decreto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che doveva essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Presidente, vorrei sollecitare anch'io

fu un voto di fiducia al Governo Prodi che di lì a poco cadde. Attraverso la perenzione amministrativa da sette a tre anni, Padoa-Schioppa è stato capace di far sparire 27 miliardi di debiti dello Stato, migliorando in apparenza il rapporto tra *deficit*

porre in essere per rimediare a questo disastro. Infatti, se anche alcuni di quei miliardi non erano veri e propri debiti, ma finanziamenti assegnati ai vari Ministeri che nei sette anni non erano stati spesi,

di sollecitare il Ministro competente a venire in Aula a dirci come intende agire per risolvere i problemi di tanti creditori dello Stato. Uno Stato che non paga i propri debiti non è uno Stato credibile.

L'ordine del giorno reca la discussione della relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sui rischi per l'efficienza dei Servizi di informazione per la sicurezza derivanti dall'acquisizione e mancata distruzione di dati sensibili per la sicurezza della Repubblica Secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, dopo l'intervento del senatore Rutelli si aprirà la discussione, per la quale ciascun Gruppo dispone di 20 minuti.

il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ho l'onore di presiedere, ha compiuto un lavoro intenso, responsabile e produttivo su una materia di estrema delicatezza. Un lavoro intenso, perché in appena 36 giorni dalla data di ricezione dei primi documenti da noi richiesti alla procura generale di Catanzaro, abbiamo svolto 12 audizioni, esaminato migliaia di pagine (con le modalità di riservatezza che comportano per i membri del COPASIR di svolgere il loro impegno esclusivamente nei locali del Comitato) e trasmesso la nostra relazione alle Camere. Un lavoro responsabile, perché la relazione al Parlamento sui rischi per l'efficienza dei Servizi di informazione per la sicurezza derivanti dall'acquisizione e mancata distruzione di dati sensibili per la sicurezza della Repubblica è stata approvata all'unanimità con grande senso istituzionale, nonostante questa materia abbia incrociato vivaci discussioni pubbliche e scottanti argomenti di attualità legislativa, a partire dal disegno di legge in materia di intercettazioni. È stato, infine, un lavoro produttivo. Sento il dovere di ringraziare i miei nove colleghi - quattro senatori, a partire dal vice presidente Esposito, e cinque deputati - perché dal nostro impegno collegiale sono derivate iniziative di collaborazione con altre autorevoli istituzioni e proposte che l'Assemblea del Senato può iniziare a valutare a partire da questa seduta. Ho trasmesso al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati una comunicazione riguardante alcuni ulteriori rilevanti profili emersi nel corso dei nostri lavori che è stata illustrata ed esaminata in un'apposita Conferenza dei Capigruppo a Montecitorio il 26 febbraio scorso. Abbiamo trasmesso all'Autorità delegata al Sistema di informazione per la sicurezza, come richiesto, i documenti necessari perché il Presidente del Consiglio possa valutare la sussistenza dei presupposti per l'apposizione e la tutela del segreto di Stato. Abbiamo trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, su sua richiesta, in spirito di collaborazione istituzionale e con il vincolo di segretezza proprio degli atti del COPASIR,

dallo scorso 13 febbraio. Essa descrive i lavori svolti dal Comitato; affronta analiticamente, seppur garantendo la riservatezza dei nomi dei funzionari dei Servizi, i fatti riguardanti l'acquisizione dei dati di traffico ed altre questioni che toccano l'attività dell'*intelligence*; riassume i dati numerici acquisiti. Nella premessa e nelle conclusioni, la relazione inquadra una vicenda che non può essere assolutamente definita di ordinaria amministrazione ed avanza alcune proposte di ordine normativo ed organizzativo. Cercherò quest'oggi di precisarle meglio, anche sviluppando alcuni temi contenuti nella comunicazione resa ai Presidenti delle Camere, concernenti alcune questioni rilevanti non strettamente riferibili alle competenze del Comitato, ma di sicuro interesse del Parlamento. Signor Presidente, si tratta di una vicenda di enorme rilievo per le istituzioni democratiche. Sia chiaro: il Comitato non ha inteso esprimere giudizi sull'attività della procura di Catanzaro a proposito dei due procedimenti denominati Poseidone e Why not?. Abbiamo espresso rispetto nei confronti di indagini giudiziarie che si sono svolte in contesti delicati. Tocca agli uffici giudiziari valutare alcune dichiarazioni che abbiamo raccolto, anche presso il Comitato, contenenti una lettura critica delle ragioni che avrebbero portato all'avocazione di quelle indagini. Il rilievo istituzionale di questa vicenda riguarda, a mio avviso, quattro punti principali. In primo luogo, l'acquisizione di dati estremamente sensibili riguardanti l'ex direttore del SISMI, il generale Nicolò Pollari. Sono state individuate le sue conversazioni telefoniche e la lista dei suoi interlocutori per 20 mesi del suo mandato di Capo del Servizio segreto militare. Attraverso i tabulati, che includevano queste informazioni, è stata verosimilmente tracciato - abbiamo acquisito elementi in questo senso - il percorso dei suoi spostamenti per lo stesso periodo di tempo: 10 marzo 2005 - 15 dicembre 2006. Lo stesso è avvenuto per due stretti congiunti del generale Pollari. È certo che questa attività sia stata compiuta nella piena consapevolezza dell'identità delle persone di cui sono stati acquisiti i tabulati di traffico telefonico. Non è stato illustrato alcun legame tra questa attività invasiva e l'indagine giudiziaria che, com'è noto, riguardava presunte malversazioni e corruzioni relative a fondi comunitari e regionali in Calabria. luogo, in base ai dati a noi noti, sono stati acquisiti i tabulati del traffico telefonico di altre 17 utenze mobili e 11 utenze fisse utilizzate da appartenenti ai Servizi, per i quali l'accertamento è stato parimenti invasivo. Il coinvolgimento nelle indagini giudiziarie di esponenti dei Servizi è stato più volte evocato anche in dichiarazioni pubbliche. Il Comitato non ha acquisito su questo alcuna informazione significativa, nonostante le puntuali e ripetute richieste avanzate nel corso delle audizioni: di ciò il Comitato non può che essere profondamente insoddisfatto, poiché suo compito istituzionale è proprio quello di controllare la correttezza dell'operato dei Servizi ed è quindi anche presso il Comitato che questi aspetti di coinvolgimento - se effettivamente sussistenti - avrebbero dovuto essere rappresentati. Ricordo che l'articolo 31, comma 4, della legge n. 124 del 2007 stabilisce che tutti i soggetti auditi dal Comitato sono tenuti a riferire con lealtà e completezza le informazioni in loro possesso concernenti le materie d'interesse del Comitato luogo, la tecnica d'indagine sviluppata dal consulente cui il pubblico ministero di Catanzaro ha delegato lo svolgimento degli accertamenti ha portato ad acquisire un numero impressionante di dati: secondo un'informazione riferita al Comitato dal ROS dei Carabinieri, si tratterebbe di una cifra oscillante tra i 14 e i 18 milioni di righe di traffico telefonico. Tra questi dati, sono state certamente acquisite informazioni sensibili, per le quali non si è potuta conoscere, signor Presidente, la necessità o l'utilità per le indagini: questo non è, per altro, nostro compito; non è compito del Comitato parlamentare. Emblematico, tuttavia, è stato il caso del procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, del quale sono stati acquisiti i tabulati di 24 mesi di traffico telefonico, nonostante lo stesso pubblico ministero responsabile delle indagini abbia dichiarato di essere all'oscuro di questa attività svolta dal suo consulente. Ogni cittadino italiano può ben comprendere la delicatezza della disponibilità di queste informazioni: può comprenderlo anche chi magari sia meno sensibile alla tutela dei dati, protetti dalla legge, riportati nei tabulati di almeno 13 parlamentari, Ministri e Sottosegretari di Stato, nonché delle utenze - e qui parliamo di utenze, lo sottolineo - di 14 numeri riferiti alla Presidenza della Repubblica e di 52 utenze fisse e mobili del Consiglio superiore della magistratura. Alcuni giorni prima dell'inizio di un'ispezione disposta dal Ministero della giustizia, sono stati acquisiti i tabulati del capo degli ispettori capo degli ispettori e quelli riferiti ad una lunghissima serie di Ministeri, uffici giudiziari, corpi dello Stato, luogo, questa banca dati, benché largamente non utilizzata per lo svolgimento delle indagini, risulta oggi nella disponibilità in base alle informazioni raccolte dal Comitato, che comunque non possiamo definire esaustive - di tre distinti uffici giudiziari (le procure della Repubblica di Catanzaro, di Salerno e di Roma) e del consulente, dottor Gioacchino Genchi, che, per quanto risulta e in base a ciò che lui stesso ha dichiarato, non ha distrutto i dati in proprio possesso. Signor Presidente, nella sede autorevole dell'Aula del Senato, vorrei ora tradurre le acquisizioni che ho appena riassunto (rimando per il resto al complesso della relazione) in una serie di osservazioni puntuali.

che non hanno una preparazione tecnica in materia (ciò che mediamente riguarda i parlamentari, non meno che i cittadini italiani), che non è affatto vero che la disponibilità dei tabulati di traffico telefonico sia meno delicata e rilevante di quella delle intercettazioni telefoniche. Al contrario, è estremamente penetrante la capacità di disporre dell'intero sviluppo di tutti i contatti telefonici di una persona in un arco di 24 mesi (a che ora, quanto a lungo, quante volte la persona parla con tutti i propri interlocutori) e di combinare queste informazioni con la localizzazione, nello stesso periodo di tempo, resa possibile nei tabulati grazie alle celle che coprono la rete telefonica mobile in tutto il territorio e nelle aree urbane con un'approssimazione di circa 150 metri. Si tratta di un vero e proprio pedinamento elettronico sistematico. Nel caso di funzionari dei Servizi di informazione per la sicurezza e di magistrati dell'Antimafia (numerosi dei quali sono presentano una delicatezza tutto particolare. Va attentamente valutato il criterio di delega totale a svolgere, nei fatti, un'attività di investigazione e di polizia giudiziaria ad un consulente privato. Ancorché si sia trattato di un vice questore della polizia di Stato in prolungato permesso sindacale, si è provveduto ad attribuirgli incarichi professionali retribuiti a beneficio di una società privata da lui controllata. Moltiplicando tale attività per le decine di incarichi assegnati da diversi uffici giudiziari, essa ha fatturato diversi milioni di euro. Non è chiaro perché le molteplici strutture tecniche dello Stato siano state spogliate di tali attività e perché siano state sostenute tali spese (cui vanno aggiunti i molti milioni di euro all'anno per le copiose prestazioni fornite al consulente dalle società telefoniche nell'ambito delle diverse inchieste e poste a carico dei singoli uffici giudiziari). Non si hanno garanzie di una conservazione protetta e, alla fine, della distruzione dei dati sensibili, il che, signor Presidente, è intollerabile. Sarebbe come se i dati acquisiti nel corso di indagini basate sul DNA restassero in possesso dei consulenti tecnici che hanno compiuto le analisi. Il Garante della *privacy* ha già emanato direttive restrittive sulle modalità operative di varie figure di consulenti che trattano dato sensibili. È evidente la criticità nel caso di possibili incroci di dati anche tra diverse indagini. Più in generale, c'è da chiedersi se nelle istituzioni competenti vi sia adeguata consapevolezza della necessità di ordinare la tempestiva e certa distruzione dei dati sensibili e perché si sia registrata una tanto insufficiente collaborazione tra organi dello Stato, non fosse altro - per fornire un esempio che è alla base degli accertamenti compiuti dal COPASIR nel suggerire all'Autorità delegata di mettere in sicurezza i dati sensibili riferiti al capo del Servizio segreto militare del nostro Paese. Resta misteriosa la ragione di tutta una serie di acquisizioni di dati. Il nostro Comitato agisce - come sanno i colleghi - in base alla legge n. 124 del 2007, nata alla luce dell'esigenza di una più severa tutela della sicurezza della Repubblica scaturita dalla vicenda della formazione di archivi e *dossier* presso la *security* di Telecom, anche attraverso collaborazioni e complicità Noi operiamo, signor Presidente, in base all'esigenza di controllare la correttezza e la probità di quella speciale, preziosa funzione che è l'*intelligence*. Ed avvertiamo anche il dovere di vigilare perché essa non sia resa vulnerabile attraverso comportamenti pericolosi, come risulta ben chiaro - mi auguro - dal lavoro che abbiamo svolto. Ebbene: non è stato indicato alcun legame tra l'indagine e l'acquisizione, da parte della procura di Catanzaro, dei dati di traffico telefonico proprio dei principali protagonisti della vicenda Telecom. Concludo, colleghi senatori, ribadendo che il COPASIR proseguirà nel suo lavoro di acquisizione di elementi connessi ai propri compiti istituzionali nell'ambito delle questioni richiamate nella nostra relazione. Procede intanto l'indagine aperta presso la procura della Repubblica di Roma che ha disposto lo sviluppo della banca dati ricevuta da Catanzaro (poco più di 70 posizioni erano state compiutamente sviluppate, in base alle informazioni trasmesse al COPASIR, sulle 1.402 che risultavano acquisite). Nelle forme, nei tempi e nei modi che il Parlamento deciderà di stabilire, vi sono alcune questioni che meritano un approfondimento e, auspicabilmente, interventi normativi. L'efficacia e la correttezza dei rapporti tra il pubblico ministero ed il consulente di cui esso decida di avvalersi, al fine di evitare che alcune funzioni proprie del pubblico ministero, quale tutore della legalità delle indagini (e per questo parte integrante dell'ordine giudiziario), signor ministro Alfano, siano devolute senza effettivi controlli. La necessità di non sostituire, attribuendole a soggetti privati, le funzioni della polizia giudiziaria (specie per alcune tipologie di consulenza). Il rafforzamento delle risorse e delle capacità operative delle forze di polizia, chiamate a trattare e conservare dati sensibili per la *privacy* dei cittadini. Il miglioramento delle garanzie nell'acquisizione ed utilizzo dei tabulati di traffico telefonico, specialmente nella certezza della loro distruzione al termine delle indagini. La verifica dell'esistenza di archivi informatici, frutto di indagini svolte negli anni passati e della loro disponibilità da parte di privati; la loro sicura distruzione e la sanzionabilità effettiva nel caso di un loro illegittimo utilizzo; la tracciabilità di questi dati nei casi di future indagini. Il rafforzamento del sistema delle garanzie: dalla non ulteriore accessibilità dei dati sensibili acquisiti alla creazione di sistemi effettivamente impermeabili. Il miglioramento delle garanzie funzionali necessarie per le attività dei Servizi di informazione - so che il Governo sta meditando una iniziativa legislativa - secondo il giusto equilibrio

normativa che il Parlamento può valutare, alla luce di queste riflessioni, nelle modalità che riterrà più opportuno di avviare e di intraprendere. Infine, la definizione di un sistema che consenta di associare in modo inequivoco un'utenza telefonica ad un membro del Parlamento, evitando al contempo ogni abuso delle prerogative parlamentari. contributo, signor Presidente. Credo spetti al Senato ed alla Camera, nella pienezza della sovranità propria del Parlamento, valutare quali iniziative assumere alla luce delle riflessioni che ho portato all'attenzione della nostra Assemblea, e delle considerazioni che saranno svolte dai colleghi che interverranno nel dibattito. La ringrazio, signor Presidente, e ringrazio i colleghi senatori Presidente Rutelli, sono io che ringrazio lei e l'organismo da lei presieduto per la la saggezza e l'altissimo senso di responsabilità con cui sono state condotte le audizioni e la gestione di questa delicatissima vicenda. inutile nascondere, anche alla luce della relazione che avete ascoltato personalmente dal presidente Rutelli, che ci troviamo dinanzi ad una vicenda estremamente emblematica, piena di risvolti delicatissimi che hanno toccato elementi e soggetti sensibili delle nostre istituzioni e del nostro Paese. Al di là dell'avere sfiorato anche la *privacy* di alcuni parlamentari, il contesto è molto più articolato ed è estremamente inquietante. Posso assicurarvi, per quanto possa dichiarare nella logica del riserbo personale che mi compete, che questa Presidenza si è tenuta sempre in stretto contatto con la Presidenza della Camera e con la Presidenza del COPASIR, la la quale ha avvertito il dovere istituzionale di informare periodicamente sia il sottoscritto che il presidente Fini, e di questo la ringraziamo. Abbiamo anche avuto opportuni contatti epistolari con alcuni organi giudiziari cui è stata devoluta la trattazione della materia.

Mi auguro che a ciò si provveda a tutela non soltanto dei diritti costituzionalmente garantiti all'articolo 68 per i parlamentari, ma anche dei diritti inviolabili di tutti i cittadini.

il Presidente del COPASIR ha presentato, prima ai Presidenti delle Camere, come previsto dalla legge istitutiva, e quindi, su nostra richiesta, al Parlamento. Ciò che emerge dalla relazione puntuale del presidente Rutelli dà uno spaccato gravissimo della situazione. dà uno spaccato gravissimo della situazione. Ad esempio, con riferimento alla questione degli archivi e delle banche dati abbiamo oggi in Italia una legge, quella di riforma dei Servizi segreti, che affida al Comitato parlamentare, e quindi al Parlamento, il controllo e la verifica degli archivi del DIS e dei Servizi di informazione, che quindi mette al riparo da eventuali abusi che i Servizi di *intelligence* potrebbero compiere nei confronti di privati cittadini o di chi svolge incarichi pubblici e quant'altro. Abbiamo una legge che garantisce il cittadino dagli eventuali abusi che i Servizi di informazione possono perpetrare; non disponiamo però di una disciplina compiuta che garantisca al cittadino di essere tutelato rispetto a chi, per ragioni diverse, interferisce, interviene, acquisisce dati, realizza schedature

che esaminiamo oggi la relazione del COPASIR con riferimento alla circostanza oggettiva che nell'ambito di una determinata attività di indagine, che sembra sproporzionata rispetto alle finalità per le quali è stata posta in essere, sono interessati funzionari e dirigenti dei Servizi di *intelligence*, e comunque soggetti che rappresentano ai livelli più alti funzioni estremamente delicate nel compito della prevenzione e del contrasto al crimine organizzato. Credo però che l'attività del Comitato parlamentare e di quest'Aula non possa e non debba essere limitata solo ed esclusivamente ad un esame e ad una verifica, così come non lo può essere l'attività che svolge, in maniera egregia,

e di cittadini che svolgono funzioni pubbliche con i fini più diversi e senza un adeguato controllo da parte dello Stato. Proprio per questa ragione

di natura criminale alle istituzioni, coperta dal controllo parlamentare, dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e dagli strumenti che l'ordinamento predispone per garantire che la democrazia si svolga secondo regole certe, trasparenti e assolutamente non alterabili attraverso l'utilizzo, come nel caso Telecom, di forti risorse economiche per svolgere un'attività di *intelligence* parallela, che certamente non fa onore e non ha fatto onore al nostro Paese.

vi è un'attività legata non soltanto alla tradizionale attività di intercettazione illegale, che è stato dimostrato ed è dimostrato essere possibile, praticabile ed essere di fatto

era opportuno, cioè quello della intangibilità delle comunicazioni degli operatori dei Servizi di *intelligence*. Si è previsto il rimedio solo con riferimento alla opponibilità del segreto di Stato e quindi alla utilizzabilità di dati sensibili, ma la circostanza che l'attività intrusiva sia di per sé lesiva per quel tipo di attività di *intelligence* svolta oggettivamente non è contemplata

per colpire tutte quelle situazioni in cui si costruiscono banche dati abusive, che vengono utilizzate in violazione della normativa vigente. Questi poteri non possono essere esercitati solo *ex post*, cioè una volta

tribunale di Milano) un uso distorto di tali dati e notizie, che altera il regolare svolgimento della libera iniziativa imprenditoriale e di mercato, della libera attività politica e delle istituzioni, condizionandone in maniera poco trasparente e illecita il loro funzionamento. Per queste ragioni, credo che si debbano utilizzare appieno i poteri che la legge n. 124 assegna al Comitato e al Parlamento, compresa la possibilità di formulare, come ha fatto oggi il presidente Rutelli, una serie di proposte concrete, che mettano in condizioni le Commissioni e il Parlamento di lavorare con tempestività su questi temi, che sono centrali per la nostra democrazia.

I toni grevi e pesanti da lui utilizzati non trovano un'effettiva corrispondenza nel testo scritto. Vediamo di cosa si tratta. Secondo i dati che ci fornisce il Comitato, quello che doveva essere il più grande scandalo della nostra storia

trovo questo dato nella relazione, ma evidentemente qualcuno si è occupato anche di contare il numero delle righe dei tabulati). Noi sappiamo il numero dei tabulati. La grande vicenda

di persone e i cui esiti sono stati offuscati dall'enorme polverone sollevato nel mese di gennaio di quest'anno sulla vicenda Genchi e De Magistris, che ha fatto passare in seconda, terza e quarta linea la vera notizia: la conclusione delle indagini, con i gravissimi capi di imputazione che riguardano politici, portaborse di politici, segretari di politici, imprenditori, uomini pubblici e affaristi; un'enorme inchiesta su chi ha depredato la Calabria di centinaia di milioni di euro. Questo è lo scandalo su cui la procura

Leggete i nomi delle persone coinvolte, i ruoli svolti e le accuse formulate. forse più di 100 capi di imputazione - dall'associazione a delinquere, alla corruzione, al peculato, al falso, alla truffa comunitaria, all'estorsione e tanto altro

consentono di individuare il traffico telefonico che ha interessato un'utenza telefonica non riguardano il contenuto. Si tratta certamente di dati sensibili perché si sa chi viene chiamato e da chi si è chiamati, quando si è chiamati, quanto è durata la conversazione e la cella

al processo. Si sono sentite parole pesanti come abuso e situazioni inquietanti. L'articolo 270-*bis* del codice di procedura penale non tutela i tabulati degli agenti dei Servizi segreti; vengono tutelate le conversazioni. È stato proprio il Comitato

«L'ordinamento non prevede particolari garanzie per gli appartenenti ai Servizi, dato che la legge n. 124 del 2007 si limita a definire all'articolo 28 una procedura che ne tutela le comunicazioni in caso di intercettazioni, attraverso la possibilità per il Presidente del Consiglio, che deve essere obbligatoriamente informato dall'Autorità giudiziaria, di apporvi il segreto di Stato. Trattandosi di una norma speciale, non può certamente essere interpretata in modo estensivo. Al fine anche di tutelare le capacità operative dei Servizi di sicurezza, modificazioni normative appaiono quindi opportune; esse potrebbero sostanziarsi nell'estensione ai dati del traffico telefonico, che consentono di individuare anche gli spostamenti del possessore di un telefono cellulare, del regime previsto all'articolo 28 della legge n. In quella stessa pagina della relazione il senatore Rutelli, a proposito di tale vicenda, parla di «rapporto di leale collaborazione tra gli apparati dello Stato, che deve sempre essere esercitato, e instauratosi nella circostanza tra SISMI e Autorità giudiziaria Leale collaborazione tra SISMI e Autorità giudiziaria: questo è scritto nella relazione! È vero che fa impressione pensare che vengano acquisiti i tabulati riguardanti il traffico telefonico per 24 mesi. Questa, però, è la legge. Non stupiamoci del fatto che la legge preveda la conservazione del traffico telefonico documentato per 24 mesi.

che la distruzione del traffico telefonico oltre i 24 mesi potesse provocare un danno alle indagini, ma anche all'indagato. però, prevede il periodo di 24 mesi e, quindi, i provvedimenti adottati riguardarono un periodo di 24 mesi di acquisizione dei tabulati.

di ricostruzione contraddittoria in quanto la possibilità della conoscenza che quel numero telefonico appartenesse al dottor Pollari, capo dei Servizi segreti, poteva dedursi da una rubrica telefonica contenuta in un cellulare. Quindi, attraverso un processo deduttivo dovremmo arrivare alla conclusione che, con certezza,

avendo utilizzato un'altra espressione, come egli ricorderà bene: ha parlato di ricostruzione dubbiosa in merito a questa conoscenza, che sarebbe poi la parte *clou* di tutto. Infatti, per quanto riguarda gli altri due agenti dei Servizi segreti, la procedura si è svolta nella piena collaborazione tra Autorità giudiziaria e Servizi segreti: perquisizione alla presenza di Servizi segreti, cellulari sequestrati e sigillati lasciati in custodia del SISMI, nessun segreto violato. Infatti, Rutelli ha scritto nella relazione che «il direttore generale delle DIS, prefetto De Gennaro, sulla base degli elementi acquisiti dall'AISE, ha precisato che essa - cioè non si è mai configurata come tale, ma che se ne fece solo riserva nell'eventualità che le attività di polizia giudiziaria fossero contestualmente proseguite presso l'ufficio del SISMI senza una preventiva concertazione di modalità di accesso che, nella massima trasparenza, garantissero il rispetto di quanto eccedente l'ambito dell'inchiesta e coperto da segretezza. La riserva non fu esercitata, secondo ciò che è stato riferito dal Direttore generale del DIS, in quanto intercorsero immediati e diretti accordi con l'autorità giudiziaria procedente, al fine di pervenire a una soluzione concordata tesa a conciliare le esigenze di giustizia con quelle di riservatezza». Questo lei ha scritto nella relazione. Cosa ci viene a denunziare ora in quest'Aula, in toni diversi dalla relazione? Io glielo dico con la stima che le porto, presidente Rutelli. Lei è stato molto è stato molto delicato quando ha inviato la lettera ai Presidenti delle Camere, segnalando il problema dei 13 parlamentari.

Ma c'era anche lei tra quei 13 parlamentari? Così hanno scritto i giornali, così dice Genchi nelle interviste. E allora, forse, un momento di di distacco dalla vicenda sarebbe stato preferibile. Non si può indagare su una vicenda che ha per oggetto se stessi. Non si può interrogare il pubblico ministero che ha indagato

che il suo alto senso istituzionale è riuscito a creare un diaframma tra i documenti che esaminava e ciò che è il compito istituzionale. Ma si rende conto che lei in questo modo è venuto a conoscenza di atti di indagine che non doveva conoscere?

Nel momento in cui si è imbattuto nel suo numero telefonico e nel suo tabulato, avrebbe dovuto astenersi. Sarebbe stato un gesto di delicatezza che non avrebbe cambiato il suo ruolo. Io ritengo che il suo lavoro non sia stato condizionato da questo. Penso, però, che avrebbe portato al medesimo risultato, perché la stimo e ritengo che lei sia persona al di sopra di ogni sospetto. Ma, per rispetto dei ruoli, forse una sua sensibilità maggiore sarebbe stata gradita e apprezzata da tutti, a meno che non si tratti

ipotesi che lei smentisce. Alla fine, che cosa viene fuori? Che si è trattato e si tratta di un enorme polverone strumentalizzato per arrivare al risultato che si vuole. Colpire il sistema delle intercettazioni: questo è l'obiettivo che si persegue; tutti gli strumenti sono buoni per arrivare a quel risultato, privare la magistratura di questo strumento di indagine. Non regolamentare meglio l'attività della magistratura nell'utilizzo di tale strumento d'indagine, ma eliminarlo.

che, in maniera convincente, il Comitato e il presidente Rutelli hanno avanzato. Benissimo, interveniamo con le norme, cambiamo le norme che lo necessitano, regolamentiamo meglio il sistema, ma non parliamo di abusi e di situazione inquietante,

giudizio sui lavori della procura di Catanzaro, anche se inevitabilmente i riferimenti vanno a finire lì. Prendendo atto delle circostanze esposte nella relazione del COPASIR, un rapporto peraltro dettagliato ed esaustivo, si coglie una palese discrepanza tra la forma e l'oggetto del documento. gravi intorno a un paradosso di ordinaria dissennatezza; dico «ordinaria» per un Paese che fatica a diventare normale. Come definire, se non paradossale e dissennata, la vicenda incredibile, prima ancora che incresciosa, del capo degli «007» militari spiato da un collaboratore di un giudice? Mi riferisco all'ex direttore del SISMI Nicolò Pollari, con tutta la sua famiglia e con altri 14 agenti segreti. due anni è stato tallonato, intercettato, pedinato tecnologicamente da un altro segugio, consulente di un magistrato: monitoraggio eseguito senza che nei confronti del soggetto posto sotto controllo sia stata sollevata alcuna ipotesi di reato, al punto che ad oggi nessuno può fornire qualsivoglia motivazione a supporto di una così serrata e strabiliante attività investigativa. Dice bene la relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, laddove paventa preoccupazione per i rischi che si possono determinare per la credibilità delle nostre Agenzie nei loro rapporti con gli omologhi organismi di *intelligence* di altri Paesi. Si tratta di una conseguenza verosimile, poiché se informazioni *top secret* e dati sensibili sono finiti nel *dossier* di un intercettatore qualsiasi, non è un azzardo ritenere che i Servizi segreti degli Stati amici giudicheranno necessaria qualche cautela nei rapporti con agenti la cui *privacy* viene così facilmente violata. D'altro canto, temo che vicende come quelle su cui stiamo ragionando comportino qualcosa di più e di peggio del comprovato rischio per l'affidabilità della nostra *intelligence*. Si tratta di un discredito che, più in generale, ricade sulle istituzioni per quell'incapacità di rappresentare il Paese serio che i cittadini si meritano. ragioniamo di fatti che in primo luogo costituiscono una violazione della sfera privata delle persone, in altra sede c'è chi propugna, con enfasi da ultima spiaggia della giustizia, il potere assoluto di intercettazione, senza se e senza ma, cioè senza neppure la sussistenza di indizi di presunta colpevolezza a carico dell'intercettato. Chi non riconosce questa facoltà arbitraria del magistrato è - così affermano - un nemico della giustizia. la legge abbia necessità di regole certe, tanto nel campo delle intercettazioni più tradizionali quanto di quelle innovative, che sembrano essere la specialità di quel Gioacchino Genchi, il vice questore consulente del pubblico ministero Luigi De Magistris, esperto nell'applicazione di tecniche legate allo sviluppo dei tabulati delle utenze telefoniche fisse e mobili, l'ex poliziotto delle cui gesta stiamo ragionando, un virtuoso dello spionaggio in grado di applicare una sorta di radar sulla testa delle persone arrivando a tracciarne anche gli spostamenti e i contatti. Non si tratta di privare gli inquirenti degli strumenti e delle capacità professionali che possono rivelarsi preziose nella lotta al crimine. Il fatto è che strumenti possono sì rivelarsi preziosi nella lotta al crimine ma, nel caso all'oggetto, queste intercettazioni hanno visto coinvolti molti cittadini apparentemente estranei all'inchiesta giudiziaria. Tra questi vi sono anche parlamentari e soggetti che rivestono ruoli istituzionali.

Evito di leggere i numeri, già illustrati molto bene dal presidente Rutelli, ma ricordo le operazioni Why Not? e Poseidone; si arriva così al monitoraggio dei vertici del SISMI, determinando di conseguenza, come afferma la relazione, una falla nel sistema della sicurezza nazionale. Questa falla ha prodotto l'acquisizione da parte di terzi di informazioni sensibili per la sicurezza dello Stato. Sulla base di tali fatti e considerazioni appare del tutto condivisibile la richiesta di idonea normazione espressa nella relazione in particolare, l'estensione al traffico telefonico, per quanto concerne le informazioni relative agli spostamenti personali, delle misure di secretazione previste dall'articolo 28 della legge n. 124 del 2007 in caso di intercettazioni per le comunicazioni di appartenenti ai servizi di sicurezza. Quindi, riteniamo motivata e urgente anche la proposta adozione di misure utili a impedire la costituzione di banche dati ricavate da privati sulla base di attività di indagine finanziate dallo Stato. Concludendo, conveniamo poi sulla necessità di colmare la mancanza di regole relative alla distruzione dei dati personali se frutto di intercettazioni che si rivelino estranee all'indagine per cui sono stati raccolti. Sempre in materia di riservatezza, condividiamo l'opportunità di inquadrare in norme precise il ricorso al tracciamento degli spostamenti forniti dal monitoraggio tramite la telefonia mobile, che viene giudicato non meno invasivo delle intercettazioni telefoniche. Si tratta di proposte serie che, come la relazione del Comitato nel suo complesso, contrastano con la burlesca circostanza degli 007 spiati da cui prende piede questa vicenda. Soprattutto queste prese di posizione vengono a dirci, caro presidente Rutelli, che la questione intercettazione non è semplicemente affare dei magistrati, ma anche e soprattutto della politica e dei cittadini.

è quanto meno strano, forse emblematico, che ci troviamo oggi in Aula a discutere di una vicenda investigativa processuale piuttosto grave e solamente a seguito di una relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Comitato che è dovuto intervenire nella vicenda soltanto perché notizie di stampa riferivano di un coinvolgimento di personale dei servizi informativi italiani all'interno di indagini penali; Comitato che ha operato ai limiti della propria competenza, ma certamente entro tali limiti, in quanto l'organismo parlamentare deve verificare che l'attività del sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni (così recita l'articolo 30 della legge n. 124 del 2007). Dico ai limiti della propria competenza proprio perché, storicamente e istituzionalmente, questo Comitato non ha il compito di tutelare dalle indagini penali gli uomini dei nostri Servizi segreti, i quali, di fatto e in diritto, anche in questa vicenda, erano e sarebbero in grado di tutelarsi da soli sia personalmente che come apparato, grazie anche alle novità legislative sulle garanzie funzionali introdotte con la legge 124 dell'agosto 2007. Il Comitato è stato costituito per altri motivi: come organo di controllo, espressione del Parlamento, sulle attività dei servizi segreti e sulla gestione del segreto di Stato. Il Comitato deve verificare che il comportamento degli appartenenti al sistema di sicurezza sia rispettoso delle regole, di tutte le regole del nostro sistema democratico e questo va sottolineato oggi, nel giorno in cui la Corte costituzionale sta decidendo in ordine ad un delicatissimo conflitto di attribuzioni tra magistratura e Governo relativamente al caso Abu Omar. Preciso questo in quanto, nel testo della relazione, mi è sembrato di ravvisare una forse inconsapevole preoccupazione di dover tutelare da ogni tipo di indagine gli uomini dei nostri Servizi segreti, addirittura oltre i timori espressi dai vertici dei Servizi segreti (si veda in particolare quanto sostenuto dal direttore dell'AISE, ex SISMI). Servizi che, anzi, per la parte di loro competenza, pare abbiano considerato di modesta valenza l'intera vicenda cosiddetta Genchi beccandosi, tra l'altro, dal Comitato parlamentare un'accusa di - letteralmente - insufficiente percezione e di sottovalutazione dei rischi. A mio giudizio, per la parte e per i fatti di competenza dei nostri Servizi segreti, ritengo che debba essere condivisa la valutazione maturata dagli stessi Servizi proprio perché essi sono sicuramente in grado di gestire situazioni di tal genere, di fatto e in diritto, con gli strumenti già previsti dalla legge, ma con due riserve. è determinata dal fatto che gli atti finora esaminati dal COPASIR sono di certo una parte ancora limitata dell'intera indagine; la seconda è costituita dal fatto che incomprensibilmente - e bisognerà chiederne conto nonostante reiterate richieste, come sostiene il Comitato parlamentare, il ROS dei Carabinieri non ha trasmesso al Comitato stesso i dati completi su supporto informatico, rimasti, peraltro, in possesso, oltre che della Polizia giudiziaria e della magistratura, anche del consulente Genchi (per quale motivo?). Precisato tutto ciò, rimangono fortissime perplessità e pesanti dubbi sulla vicenda investigativa che ha riguardato decine di rappresentanti delle istituzioni di ogni ordine e grado. a parte le anomalie particolarmente significative di carattere istituzionale comunicate dal COPASIR ai Presidenti delle due Camere (anche se non si spiega quali sono se si tratta di violazioni dell'articolo 34 della legge n. 124; e se sì, per quale motivo l'informativa non viene trasmessa anche al Presidente del Consiglio dei ministri?), a parte queste anomalie particolarmente significative - così denominate dal COPASIR - non vi è dubbio che l'intera vicenda sia particolarmente grave, perché fortemente invasiva della sfera privata di cittadini normali e di altre autorità e soprattutto perché non coinvolti formalmente in alcuna indagine e in alcuna accusa. vicenda, come dicevo, ma non per aver coinvolto qualche uomo dei nostri Servizi segreti, quanto piuttosto per la disinvolta gestione di dati e informazioni molto, molto sensibili: e si tratta di una gestione posta in essere in occasione di un'indagine giudiziaria penale.

di informazioni complete e più precise su quanto è successo, secondo quanto segnalato al Parlamento dal COPASIR, consiglia un minimo di cautela, in attesa di riscontri più adeguati, sia sul contenuto delle indagini sia sul coinvolgimento di soggetti istituzionali. Di certo, però, si rimane allibiti, istituzionalmente, di fronte all'uso assolutamente abnorme che è stato fatto di norme e strumenti investigativi, così come dello spazio e dei poteri concessi ad un consulente tecnico. Ne è scaturita la gestione, da parte di un consulente privato, di dati sensibili e archivi informatici a dismisura; gestione che risulta del tutto ingiustificata dal punto di vista istituzionale e non consentita da alcuna normativa al termine delle indagini: forse è il caso di intervenire, anche legislativamente, in maniera precisa e più articolata in materia di banche dati, soprattutto se gestite da privati, o comunque di interessare della vicenda in modo più specifico l'Autorità garante della*privacy*, sulla scia, peraltro, delle sue linee guida, già adottate *ante litteram* il 26 giugno 2008. Attenzione, però, a non strumentalizzare la vicenda e a non utilizzarla per proporre limitazioni dei poteri di indagine delle forze di polizia e della magistratura, soprattutto in materia di intercettazioni, che non c'entrano assolutamente nulla con il comportamento del consulente Genchi che trattava soltanto di tabulati.

di indagine, che va assolutamente stroncato, con gli strumenti penali e disciplinari già esistenti, nell'interesse stesso delle istituzioni e del nostro sistema democratico, senza però coinvolgere in questa necessaria opera di chiarezza, trasparenza e pulizia, istituti e mezzi investigativi assolutamente indispensabili. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, la relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica al nostro esame apre uno squarcio su una vicenda a dir poco inquietante. inquietante per i rischi indotti al nostro sistema di informazione per la sicurezza, in quanto, coinvolgendo anche il personale operante nei Servizi, pone un serio problema sulla credibilità stessa dei Servizi. inquietante per il coinvolgimento, nelle inchieste giudiziarie condotte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, di molti cittadini estranei alle inchieste, tra i quali anche parlamentari e soggetti che rivestono ruoli istituzionali evocando i sinistri spettri dello Stato poliziesco (il «grande fratello» di orwelliana memoria). inquietante per l'immagine che ha dato sul piano internazione dei nostri Servizi segreti con danni inimmaginabili sulla loro credibilità. A tal proposito condividiamo la preoccupazione espressa con forza dal Comitato nella sua relazione. La formazione di vere e proprie banche dati, ricavate da indagini finanziate dallo Stato, al di fuori di ogni controllo e realizzate da un uomo dello Stato, un vice questore aggiunto della Polizia non già però nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ma come consulente privato, appare un *vulnus* gravissimo alla sicurezza della Repubblica, a quel rapporto di leale collaborazione tra apparati e organi dello Stato che dovrebbe essere la pietra su cui si regge questo Paese: un vero e proprio attentato democratico. Ancora una volta questa vicenda ci fa riflettere sull'urgente necessità di porre mano, da un lato, ad una riforma della giustizia che eviti il ripetersi di fatti analoghi, con pubblici ministeri legati a filo doppio a consulenti privati spregiudicati, strapagati e utilizzati per lo svolgimento di accertamenti istruttori delicati, e, dall'altro, ad una riforma del tema delle intercettazioni telefoniche e del sistema legale delle intercettazioni per garantire almeno un livello minimo di sicurezza e riservatezza. Le intercettazioni telefoniche sono uno strumento di indagine invasivo della sfera individuale della persona umana e l'invasività del mezzo diventa odiosa e ripugnante se piegata a finalità che nulla hanno a che vedere con le finalità di giustizia e con i fatti oggetto delle indagini. Sappiamo che le intercettazioni telefoniche sono indispensabili per poter sperare non già di eliminare, ma di fronteggiare ed in certa misura contenere fenomeni criminosi come quelli della criminalità organizzata. Marcello Maddalena - lasciatemi citare il pensiero di un noto magistrato - nel marzo del 1996 scriveva che le intercettazioni telefoniche «sono un male, ma un male necessario». Proprio perché sono un male, seppur necessario, occorre circondare l'uso di questo strumento devastante di una serie di garanzie potenziate ed estese rispetto a quelle oggi vigenti. E soprattutto occorre evitare che tale strumento investigativo possa essere utilizzato da consulenti privati, magari in aspettativa sindacale, anziché da strutture delle forze di polizia. Il caso Genchi è solo la punta dell'*iceberg* e dobbiamo cogliere l'opportunità della discussione dell'ampia relazione del Comitato (che ringraziamo per la sua attività) per ribadire con fermezza che questo Paese non può trasformarsi in una immensa cloaca collettiva in cui i veri interessi della giustizia non c'entrano per nulla e, anzi, hanno tutto da rimetterci, soprattutto quando dietro le intercettazioni, e la diffusione del loro contenuto, vi è non tanto un interesse di giustizia o di democrazia, bensì un interesse specifico allo *scoop* giornalistico, anche a danno della reputazione altrui. Può darsi che le riforme che abbiamo indicato come necessarie comportino il parziale sacrificio di qualche «sacro principio», ma di sacri principi si può anche morire per asfissia.

è perché ce ne offre lo spunto concretissimo la relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che il suo Presidente, senatore Rutelli, ci ha illustrato ha ad oggetto le modalità di svolgimento e gli sviluppi di due note inchieste della Procura della Repubblica di Catanzaro. Ritengo che la relazione esponga dei fatti di assoluta gravità e credo che il Senato abbia il dovere di esprimersi con grande franchezza e chiarezza, come hanno fatto sinora i senatori intervenuti, e senza reticenze. So di ripetere qualcosa di ben noto a tutti noi, ma il Senato non è un tribunale e non abbiamo il potere di attribuire patenti di innocenza, di colpevolezza o di interferire sul lavoro della magistratura che tutti vogliamo libera ed indipendente. Abbiamo però il dovere di esprimere giudizi politici e di assumere le conseguenti iniziative parlamentari. La relazione ha sottoposto all'attenzione del Parlamento delle anomalie numerose e molto rilevanti e non possiamo archiviarle come il mero frutto di una comprensibile difficoltà di una indagine complessa e, all'origine, non definita. Non voglio ripetere nel dettaglio quanto già i colleghi intervenuti e il presidente Rutelli hanno già ampiamente hanno già ampiamente illustrato. Tuttavia, sinteticamente, debbo ricordare - affinché il ragionamento che vorrei svolgere possa funzionare - che è vero, come ricordava il senatore Li Gotti, che l'indagine ha a che fare con circa 1500 tabulati di traffico telefonico, ma è anche vero che le acquisizioni anagrafiche che sono state disposte nell'ambito dell'indagine riguardano circa 400.000 intestatari telefonici. Non so quante siano le righe, ma circa 400.000 sono i nomi sui quali sono stati richiesti particolari sull'intestazione. Naturalmente, non sfugge a nessuno di noi l'importanza che tra gli interessati a queste indagini vi fossero numerosi parlamentari, la Procura nazionale antimafia,

al fatto che, in una indagine importante, vengano richiesti tabulati o dati anagrafici anche di alte personalità dello Stato che ricoprono delle responsabilità importanti.

quando nella relazione è scritto che, riguardo a tali attività, non è stato individuato il confine tra la legittimità di accertamenti volti a perseguire attività illecite e la molto meno legittima attenzione nei confronti di situazioni totalmente estranee alle indagini, questo mi interessa e lo considero un elemento molto importante per giudicare ed esprimere un giudizio politico sui fatti che oggi siamo chiamati a a commentare in quanto descritti nella relazione. Mi interessa egualmente leggere nella relazione che un elevato numero di utenze telefoniche coinvolte nelle inchieste sono riconducibili a cittadini apparentemente estranei all'inchiesta giudiziaria. Evidentemente mi interessa anche sapere che, tra i cittadini estranei all'inchiesta giudiziaria, vi fossero dei parlamentari e dei soggetti che rivestono ruoli istituzionali. Questa mi sembra l'asse principale delle indagini di Catanzaro. Questo mi sembra il suo senso sintetico, al quale voglio aggiungere, perché può essere molto influente sull'opinione che dobbiamo esprimere sulla relazione, altri due elementi molto importanti. Il primo è che al Comitato sono stati trasmessi dati incompleti. Nonostante i dati trasmessi al Comitato fossero incompleti, sappiamo per certo che l'insieme di tali dati, acquisiti dal consulente Genchi nella sua funzione di ausiliario delle indagini, costituisce una vera e propria banca dati, che potrebbe - dice il Comitato - aver assunto dimensioni comparabili, se non addirittura superiori, a quelle di banche dati delle forze di polizia. Trovo anche molto interessante e significativo che nelle diverse fasi dell'indagine, tra il magistrato De Magistris e Genchi non fosse chiaro chi decideva e chi eseguiva. Fatto sta, che, come risulta sempre dalla relazione, il consulente sembra svolgere indagini e formulare suggerimenti. e formulare suggerimenti. Fatto sta che il pubblico ministero ha firmato decreti con lunghi elenchi di numeri telefonici da lui irriscontrabili, in quanto privi dell'indicazione dell'intestatario. Voglio rilevare che il capovolgimento dei ruoli tra consulente e pubblico ministero, comunque sia, danneggia fortemente la giustizia.

per venire a conoscenza di atti giudiziari che lo riguardavano personalmente e che avrebbe dovuto astenersi dall'entrare a conoscenza di tali atti. Egli ha anche detto che il senatore Rutelli, nello scrivere al Presidenti di Camera e Senato, avrebbe omesso di indicare il nome dei parlamentari coinvolti nell'inchiesta, in quanto il suo nome era tra quelli.

le notizie che lei ha ricevuto non dovessero risultare vere, lei avrebbe il dovere, con altrettanta solennità, di riconoscerlo in Aula. Credo inoltre che dovrebbe cercare di fare in fretta questo accertamento perché lei (ed è questo

un senso d'urgenza per alcuni interventi normativi. Ne indico quattro. Il primo riguarda la necessità di subordinare l'accesso ai tabulati del traffico telefonico e telematico del personale dei Servizi di sicurezza alle stesse garanzie previste per le intercettazioni telefoniche. Questo che parifica le intercettazioni telefoniche Il secondo riguarda la necessità di sottoporre la gestione di banche dati e di archivi informatici ricavati da inchieste giudiziarie a forme di custodia definita per legge e affidata ad una autorità pubblica. Il terzo riguarda la necessità di prevedere che per le utenze telefoniche intestate ad un parlamentare sia sempre possibile garantire che lo stesso ne sia l'effettivo intestatario e l'effettivo utente. Non è tollerabile

(che l'ordinamento prevede per ben altri obiettivi) per svolgere con elevati emolumenti, da privato cittadino incaricato dal pubblico ministero ed anche attraverso società a lui riferibili, mansioni analoghe a quelle che avrebbe dovuto svolgere come pubblico dipendente.

è se l'esistenza di un amplissimo archivio informatico, costituito sulla base di discutibili disposizioni dell'autorità giudiziaria e destinato ad essere per tempi lunghissimi nella disponibilità di professionisti che da privati svolgono, *pro tempore*, funzioni pubbliche, quali il dottor Genchi e - lo voglio sottolineare - i suoi collaboratori, costituisca un fatto isolato, ovvero sia il segno, la punta emersa di un *iceberg* molto più ampio, l'indizio di un fenomeno che, nell'indifferenza generale, è andato via via dilatandosi e che consiste in una sorta di "privatizzazione" di porzioni dì attività pubbliche che le esigenze della sicurezza della Repubblica e delle garanzie dei cittadini dovrebbero sempre e in ogni caso indurre a mantenere all'interno del monopolio e del controllo dello Stato. Gli indizi della "privatizzazione" di pezzi del sistema di sicurezza del nostro Paese sono molto evidenti. Non ho elementi sufficienti per valutare appieno l'effettivo ruolo svolto a vario titolo dai diversi protagonisti privati che ruotano intorno al sistema nazionale la relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ci ha informato che in Italia esistono sofisticate banche dati che contengono informazioni altamente sensibili.

senza che la legge preveda quale sorte debba avere il materiale da loro raccolto una volta terminata l'indagine. Non sappiamo e non siamo in grado di escludere che, oltre alla banca dati nella disponibilità del dottor Gioacchino Genchi, ve ne siano altre simili, magari anche ampiamente duplicate. In teoria potrebbe essere così. Sappiamo poi che in Italia gran parte del sistema delle intercettazioni telefoniche viene affidato in *outsourcing* dall'amministrazione della giustizia ad operatori telefonici privati. Sappiamo che è un sistema molto costoso e che in passato vi sono stati operatori che hanno abusato delle funzioni e della strumentazione che lo Stato ha loro affidato. Sappiamo che grandi aziende italiane hanno creato strutture interne di *security* di dimensioni molto consistenti, con *budget* rilevanti, con ampiezza di funzioni, alle dirette dipendenze del capo azienda. Nelle prossime settimane si aprirà a Milano un processo che considero molto importante, che vede coinvolta quella che dal 2001 era la struttura di *security* della Pirelli, poi trasferitasi in Telecom, risultata talmente implicata in operazioni di dossieraggio illegale da rendere conveniente a Telecom e a Pirelli disporre congrui risarcimenti a favore dei dipendenti delle due aziende oggetto delle attenzioni della *security*. Non sto forzando la lettura degli avvenimenti e dei comportamenti. In assenza di adeguate spiegazioni, tra l'archivio Genchi, l'*outsourcing* delle intercettazioni e la *security* di Pirelli-Telecom potrebbero esserci legami sottili, forse rivelatori. Rivelatore potrebbe essere, per esempio, la presenza non spiegata, tra il materiale acquisito nell'ambito delle inchieste di Catanzaro, di documentazione relativa ai nominativi di Tavaroli, Ghioni, Bove e Mancini, quest'ultimo dipendente del SISMI. La relazione del Comitato ha accertato che non sono chiare le ragioni per le quali ciò è avvenuto. Così come sarebbe singolare, Presidente, se dovesse risultare corrispondente al vero che, nel 2002, un signore con lo stesso cognome del dottor Gioacchino Genchi, il dottor Sergio Genchi, in contatto con Tavaroli, all'epoca dirigente della *security* di Pirelli, abbia collaborato con Telecom all'avvio delle trattative per la vendita di un pacchetto di azioni di Telekom Serbia ad una società di Stato serba. Sono coincidenze molto singolari, che il Parlamento ha il diritto sottolineo, il diritto - che gli vengano chiarite. Signor Presidente, è finita la guerra fredda, ma non è venuto meno il bisogno degli Stati, e del nostro Stato in modo particolare, di di disporre di Servizi di informazione e di sicurezza. Anzi, ne abbiamo forse più bisogno oggi di allora. L'emergere di potenze medie e grandi regionali, la globalizzazione, le tensioni economiche, la criminalità internazionale, tutti motivi che rendono necessario al nostro Paese di disporre di Servizi di sicurezza leali ed efficienti. Il Senato deve sapere che questo obiettivo non può essere raggiunto attraverso forme più o meno striscianti di "privatizzazione" dei sistemi di sicurezza. Solo il rafforzamento delle istituzioni pubbliche può garantire la sicurezza della Repubblica e, con essa, la libertà e i diritti dei cittadini. Signori senatori, si sottopongano pure le istituzioni pubbliche a tutte le verifiche e a tutti i controlli che sono considerati necessari per garantire al Paese la loro lealtà, ma non abdichiamo, a favore di entità private, al principio democratico che attribuisce allo Stato, e solo allo Stato, il monopolio della forza, della giustizia e della sicurezza.

Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, fin dal primo momento in cui sono apparse chiare le dimensioni della vicenda che il presidente Rutelli ha affrontato nella sua relazione, abbiamo voluto che ad occuparsene fosse il Parlamento nella sua interezza, consapevoli delle competenze e delle prerogative che sono assegnate al COPASIR e dunque anche dei loro limiti. Si è evitato di cadere nel gioco di chi, con rivelazioni vere o più probabilmente presunte, con condizionali, avrebbe voluto trasformare il Comitato in un'impropria Commissione di inchiesta. Dunque, al cospetto di acquisizioni come quelle che abbiamo ascoltato, si è giustamente deliberato di investire della questione la Presidenza delle Camere e, per quel che è di sua competenza, la procura della Repubblica. Al tempo stesso, questo di evitare che le informazioni, le congetture e le ricostruzioni fuoriuscite dall'ambito istituzionale possano, da una parte, continuare ad alimentare una discussione distorta e asimmetrica nella quale le versioni date in pasto all'opinione pubblica siano unilaterali, dettate dall'uso spregiudicato dei *mass media* a fronte di una dovuta riservatezza dei membri del COPASIR; o, dall'altra, finire in una sorta di terra di nessuno. Si è dunque avvertita l'esigenza di porre rimedio a questa situazione di oggettivo squilibrio che rischiava di inquinare il dibattito pubblico, a detrimento della verità e della consapevolezza dei cittadini. Per questo, signor Presidente del Senato, sentiamo di doverle essere grati perché, unitamente al Presidente della Camera, ha mostrato sensibilità istituzionale nei confronti di questa esigenza e con sollecitudine ha voluto convocare questa seduta. Credo che la stessa gratitudine dovrebbe essere espressa - ed è stata espressa, d'altra parte - dai colleghi dell'opposizione, che oggi hanno avuto anche la possibilità di rimediare all'errore di chi, tra le loro fila, alle prime avvisaglie di ciò di cui al COPASIR si stava man mano acquistando contezza, ha tentato di far credere che da parte del Governo e della maggioranza si volesse approfittare di un caso, gonfiandolo a dismisura, al solo scopo di perpetrare un colpo di mano sulla normativa che disciplina le intercettazioni telefoniche. La relazione del presidente Rutelli fa evidentemente strame di ogni insinuazione, e autorizza a sperare che da ciò che abbiamo ascoltato la stessa opposizione possa ricavare elementi di allarme per la libertà dei cittadini, per la sicurezza dello Stato e per il funzionamento stesso dell'ordine giudiziario, e giungere a condividere la necessità di interventi normativi volti a rafforzare un sistema di garanzie evidentemente fallace. Delle intercettazioni telefoniche parleremo più avanti.

che gli stessi limiti e le stesse garanzie relative all'utilizzo e al controllo degli strumenti di comunicazione siano estesi anche alle anagrafiche tributarie e ai tabulati. Dalla discussione di questa sera potrà provenire, dunque, un contributo al dibattito più ampio su cosa significhi nel nostro Paese il rispetto dei diritti fondamentali della persona e sulla necessità che la tutela della legalità e lo Stato di diritto non vengano mai posti in contrapposizione. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, non è infatti sufficiente chiedersi se ci troviamo di fronte a un caso di comportamento delittuoso, di assoluta violazione della legge, rispetto al quale l'apparato pubblico possa attivare i propri anticorpi, per così dire "naturali", perseguendo i responsabili e ripristinando la legalità. Preferiamo che a occuparsi di questi aspetti sia l'autorità giudiziaria. La rilevanza politica della vicenda di cui stiamo discutendo è data dal fatto che tutto ciò sia potuto avvenire insinuandosi persino tra le maglie delle procedure, alternando probabili abusi con pratiche *border line* e finanche formalmente regolari, messe in atto nel migliore dei casi con la colpevole distrazione dell'autorità giudiziaria che quelle pratiche ha avallato o comunque ha formalmente autorizzato. tutto questo - lo ripetiamo - pone evidenti problemi in ordine alla sicurezza dello Stato, alla libertà individuale dei cittadini e allo stesso corretto funzionamento del sistema giudiziario. Che cosa è accaduto? Lo abbiamo già sentito, ma è bene ripeterlo: nell'ambito di due procedimenti penali aperti presso la Procura della Repubblica di Catanzaro un consulente privato, individuato e "arruolato" da un pubblico ministero (per di più poliziotto in aspettativa sindacale da circa un decennio), ha chiesto e ottenuto dallo stesso magistrato l'autorizzazione all'acquisizione di un numero abnorme di intestatari anagrafici, anagrafici, di utenze e di tabulati di traffico telefonico, relativi a una molteplicità di soggetti non coinvolti nelle indagini. Tra questi, gli accertamenti hanno consentito l'individuazione - anche questo lo ripetiamo - di dati relativi a parlamentari, ministri, magistrati, utenze della Camera e del Senato, a diversi Ministeri, alla Presidenza del Consiglio, all'Ambasciata degli Stati Uniti, al Consiglio superiore della magistratura, al segretariato generale della Presidenza della Repubblica, alla Guardia di finanza e a partiti politici. E ancora, e soprattutto, tale attività ha determinato la vulnerabilità dei nostri apparati di sicurezza attraverso l'acquisizione dei dati di traffico e dunque dei contatti e degli spostamenti di esponenti di rilievo dei Servizi, fino addirittura all'ex direttore del SISMI, generale Nicolò Pollari. È stato, dunque, compromesso e profanato l'ambito più sensibile e riservato all'interno dell'apparato che tutela la sicurezza dello Stato senza che neppure l'autorità governativa delegata a sovrintendere sull'attività di *intelligence* ne sia mai stata messa a conoscenza. Per ragioni che sfuggono, inoltre, tra l'acquisizione dei tabulati risulta anche quella relativa ad utenze - ha ragione il senatore Zanda - riconducibili a Giuliano Tavaroli, Fabio Ghioni e Adamo Bove, già responsabili o componenti della *security* di Telecom, al centro di un'altra vicenda altrettanto estesa quanto a dimensioni ma diversa perché maturata nell'ambito di un'azienda privata e, se rispondono al vero le ipotesi di accusa, di fuori delle maglie della legge tant'è vero che la magistratura è in questo caso prontamente intervenuta. Infine, attraverso accertamenti che solo all'apparenza non sembrano essere invasivi, è stata violata la *privacy* di molti cittadini non sottoposti ad indagine, a Catanzaro, ma non solo. Qualche numero aiuterà a comprendere di cosa stiamo parlando: limitatamente ai dati forniti al COPASIR da Telecom, al netto dunque delle utenze riferibili a tutti gli altri gestori telefonici, risulta che il consulente Genchi, autorizzato da 28 diversi uffici giudiziari, ha chiesto tra il 2004 ed il 2008 5.517.579 anagrafiche e tra il 2002 e il 2009 24.343 tabulati; per quanto riguarda le inchieste del procuratore De Magistris "Why not?" e "Poseidone", siamo nell'ordine di oltre 2.000 tabulati e di quasi 500.000 anagrafiche. C'è da chiedersi se tutto ciò è avvenuto dietro impulso di un'autorità giudiziaria inquirente pienamente consapevole, oppure se è stato il consulente privato a guidare gli accertamenti spingendosi fino a formulare congetture e piste di indagine, con un pubblico ministero ridotto alla mera funzione notarile di autorizzare l'acquisizione elefantiaca di dati dalla dubbia pertinenza. Da quanto abbiamo appreso dalla viva voce del pubblico ministero, era il consulente a guidare di fatto le indagini attraverso le sue richieste di acquisizione. Da parte sua, al contrario, il consulente ha riferito al COPASIR che nessun atto è stato compiuto senza il pieno coinvolgimento del magistrato. Le versioni, come è evidente, si contraddicono l'una con l'altra. Non ci si può, dunque, esimere dal rilevare come nel peggiore dei casi il rappresentante dello Stato, ovvero il pubblico ministero, abbia consapevolmente preso parte all'attività del consulente; nella migliore delle ipotesi, si è reso responsabile di omesso controllo. C'è da chiedersi anche se si possa continuare a tollerare che l'autorità giudiziaria, fatta salva la possibilità di ricorrere a professionalità esterne per specifici accertamenti soprattutto di natura tecnica, deleghi a privati attività così delicate per la libertà dei cittadini, che pure la polizia giudiziaria sarebbe perfettamente attrezzata per svolgere. Si tratta di un interrogativo impellente perché, oltre alla fase dell'accertamento, investe anche il momento della conservazione di dati così sensibili, che da strumenti di indagine possono diventare arma di ricatto nei confronti di qualunque cittadino. È evidente, infatti, che l'attività di cui ci occupiamo questa sera sia stata compiuta in aperto contrasto con il provvedimento adottato nel giugno scorso dal Garante della *privacy* che riguarda i consulenti dell'autorità giudiziaria e chiarisce che il materiale di indagine debba rimanere presso gli uffici di procura e possa essere trattenuto dal consulente solo se autorizzato dal pubblico ministero o se previsto da una specifica norma di legge. Lo stesso provvedimento prescrive, inoltre, che possano essere trattenuti solo i dati necessari e che da parte del consulente non possa essere compiuta alcuna ricerca di propria iniziativa. Signor Presidente, collaboratori del consulente, secondo quanto riferito dal consulente medesimo, hanno preso visione del materiale di indagine relativo alle inchieste di Catanzaro. Chi sono questi collaboratori? Chi può garantire che dei dati non siano stati fatti ulteriori usi impropri? Chi può assicurare che tabulati e anagrafiche verranno distrutti, posto che il consulente stesso ha riferito di avere trattenuto copia integrale delle sue acquisizioni? E ancora, è tollerabile in una democrazia, in uno Stato di diritto, che un privato cittadino detenga nella sua disponibilità, con la motivazione di dover forse un domani testimoniare in un processo, i tabulati telefonici, ad esempio, dell'ex capo dei servizi segreti, di parlamentari, di ministri, di magistrati e di tanti altri privati cittadini, mai neppure sfiorati dalle inchieste del dottor De Magistris? È sicuro, signor Presidente, uno Stato in cui accade una cosa del genere? È uno Stato libero? Non si tratta di un'autotutela della classe politica. Né sarà qualche irresponsabile tribuno dalla scarsa fantasia a coprire dietro l'abusata retorica della "casta" il fatto che in gioco in questa vicenda c'è la sopravvivenza stessa dello Stato di diritto. È a repentaglio la libertà dei cittadini, la sicurezza dello Stato e anche la credibilità del sistema giudiziario, se si pensa che attorno all'archivio Genchi e alle inchieste del dottor De Magistris si è consumato il gravissimo scontro tra la procura di Salerno e la procura generale di Catanzaro che tanto sconcerto ha suscitato nell'opinione pubblica e nelle più alte cariche dello Stato. Uno scontro di cui forse abbiamo ancora una conoscenza parziale e che è lecito sospettare essere ben più ampio e più profondo, se solo si pensa che fra le utenze oggetto d'interesse del consulente della procura di Catanzaro figurano quelle del procuratore nazionale antimafia, di altri magistrati antimafia, nonché del capo degli ispettori del Ministero della giustizia. Tutto questo fa pensare che vi siano dinamiche all'interno di una parte del potere giudiziario che procedono in senso opposto rispetto alle reali esigenze dei cittadini e che lo rendono un potere autoreferenziale e soggetto ad inquinamenti interni, come dimostra anche il video che Gioacchino Genchi ha pubblicato su «You tube», realizzato dal blogdi Beppe Grillo, sul quale ci soffermeremo tra breve. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, su questo tema non sarebbe onesto tentare di minimizzare. Né è possibile giocare con le parole, tentando di far credere ai cittadini che fra le intercettazioni telefoniche e l'acquisizione dei tabulati

per le persone estranee alle inchieste la ricostruzione di un mero contatto telefonico può essere ancora più lesiva di una intercettazione, perché lascia spazio alla congettura, all'insinuazione, finanche alla minaccia. Non a caso la Corte costituzionale, in riferimento all'articolo 15 della nostra Carta, ha equiparato i dati esteriori della conversazione telefonica al suo contenuto, considerando entrambi parte del patrimonio inviolabile di ogni persona in relazione a qualsiasi forma di comunicazione. Se si considera che la stessa Corte ha sentenziato l'inammissibilità in giudizio di mezzi di prova acquisiti attraverso attività compiute in violazione delle garanzie costituzionali, se ne ricava che il materiale oggi al nostro esame è di dubbia validità, anche sotto il profilo processuale. Signor Presidente, in conclusione, non posso

per occultare una sostanza fatta di delitti, di complicità, di connivenze inconfessabili. In un gioco di detto e non detto si chiamano in causa magistrati, reparti di forze dell'ordine, giornalisti, protagonisti della vita pubblica di oggi e di ieri, da Mastella a Martelli, fino allo stesso presidente del COPASIR Francesco Rutelli, cui va la nostra solidarietà. Si chiamano in causa le stragi di mafia. Noi a questo gioco non intendiamo dare spazio. per questo auspichiamo che il dibattito di questa sera possa iniziare anche a far chiarezza su questo punto, perché se le affermazioni contenute in quel filmato sono fondate, allora è necessario che intervengano gli organismi preposti. Se sono infondate, ebbene qualcuno ne deve rispondere di fronte alle autorità competenti. Per noi, signor Presidente, lo Stato di diritto e la legalità stanno dalla stessa parte. Se qualcuno tenta di abbattere il diritto fingendo di difendere la legge, sappia che non saremo mai noi a mettere in contrapposizione la dimensione formale con quella sostanziale, e non accetteremo mai di operare una scelta a favore dell'una e a discapito dall'altra. Come rappresentanti del popolo ci sono però due interrogativi ai quali non possiamo sottrarci. Dobbiamo chiederci, signor Presidente, colleghi senatori, come sia possibile che tutto ciò sia potuto accadere. E cosa fare affinché fatti come quelli che abbiamo ascoltato oggi non accadano più. È dunque auspicabile che questo dibattito non finisca stasera e che il Parlamento trovi i modi più idonei e i tempi per continuarlo.

di proposte), sia nel raccogliere alcune proposte che abbiamo avanzato e che ho riassunto nella mia introduzione, sia con altre sottolineature fatte durante il dibattito. vorrei innanzitutto portare una ferma precisazione. Il Comitato non ha ricevuto alcun tabulato né alcuna informazione di qualunque rilievo concernente alcun membro del Comitato. Nessun membro del Comitato fa parte dell'elenco dei tredici parlamentari che ho citato a proposito dell'acquisizione dei tabulati, che erano stati in un primo tempo inseriti nella relazione, come i colleghi del Comitato sanno, ma che, d'intesa con i Presidenti delle Camere, abbiamo ritenuto

e in quella sede potranno essere svolte tutte le valutazioni competenti. Alla luce di ciò, mi aspetto le scuse del senatore Li Gotti, perché la civiltà del nostro confronto parlamentare credo non dovrebbe mai indurre a dichiarazioni come quelle che ho ascoltato qui senza la necessaria verifica. A meno che lei, senatore Li Gotti, si appoggi a qualche dichiarazione comparsa su alcuni blog; deve sapere che essa è stata già perseguita con le appropriate vie legali. C'è tuttavia un piccolo motivo di soddisfazione, Presidente, perché i colleghi qui presenti del nostro Comitato sanno quanto siano difficili le nostre condizioni di lavoro: noi lavoriamo senza poter mai portare con noi i documenti; dobbiamo lavorare presso la sede del Comitato perché essi sono coperti da segretezza. In generale, cerchiamo di rispettare questa segretezza e sono molto lieto che il rappresentante dello stesso Gruppo parlamentare, per conto del quale il senatore Li Gotti ha preso la parola, e che rappresenta quel Gruppo parlamentare in seno al nostro Comitato, sia stato talmente riservato da non informare lo stesso senatore Li Gotti del fatto che gli ho appena ricordato, ossia che nessuno dei membri del Comitato rientra nei tabulati che egli ha ritenuto improvvidamente di chiamare in causa.

dati che sono agli atti nella relazione, che sono già negli atti di questa seduta oltre che nella mia introduzione ai lavori, quanto segue. Noi siamo il Comitato di controllo sull'attività dei Servizi e vorrei assicurare tutti i colleghi del fatto che quando noi ci siamo trovati, nel corso del tempo, di fronte all'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico relativi a ventotto utenze riferite ai Servizi di sicurezza italiani, abbiamo chiesto a tutte le persone ascoltate perché questo fosse avvenuto. Questo, infatti, su tutti è il nostro compito. E posso assicurare i colleghi che non abbiamo ottenuto risposta. Questo è un punto sul quale l'Aula del Senato può svolgere, a mio avviso, una riflessione aggiuntiva riguardante, precisamente, la sicurezza della Repubblica e il corretto rapporto di collaborazione tra le istituzioni. Poi, certo, quando un organismo parlamentare apprende ciò che noi abbiamo appreso e che è stampato, nelle sue linee generali, nella relazione e negli atti di questa seduta, il nostro dovere è di darne comunicazione al Parlamento. Noi siamo un organo parlamentare, come potremmo non altrimenti riferire per le vie stabilite, al Presidente del Senato, che ha dimostrato costante attenzione, così come il Presidente della Camera, e all'Assemblea, com'è avvenuto oggi, le linee fondamentali che anche nello svolgimento del dibattito avete ascoltato?

È vero che noi non siamo un organismo inquirente: non lo siamo, non abbiamo gli strumenti e non è né il nostro mandato né il nostro compito

con un'indagine riguardante ciò che il senatore Li Gotti ricordava appropriatamente, cioè un'indagine su possibili malversazioni e scandali concernenti fondi comunitari e regionali della Regione Calabria.

è quello di una Commissione di inchiesta parlamentare con i poteri propri di una Commissione di inchiesta parlamentare; infatti, abbiamo dovuto mettere in rilievo che a molte delle domande da noi rivolte a diversi soggetti istituzionali non abbiamo ottenuto sufficiente risposta e sufficiente approfondimento. Crediamo però di avere tentato di fornire al Parlamento una pagina di verità sulla base dei dati di cui disponiamo; abbiamo cercato di dare al Parlamento un contributo di verità. Sarà compito del Parlamento, del Parlamento, alla luce di questo dibattito che sarà ora concluso con l'intervento importante del Ministro della giustizia (che ringrazio anche per aver seguito interamente questa discussione), questa discussione), intraprendere le iniziative che riterrà più opportune alla luce di questa disamina complessa, delicata e tuttavia svolta in profondità e con piena coscienza dal nostro Comitato e, da questa sera, dall'intero Parlamento. *(Applausi

Signor Presidente, vorrei preliminarmente ringraziarla per aver consentito al Paese di conoscere, nella forma più alta ed istituzionale, una delicatissima vicenda che investe anche la sicurezza nazionale. Vorrei ringraziare, inoltre, il presidente Rutelli ed il COPASIR tutto per il lavoro svolto, suggellato da un voto unanime Signor Presidente, onorevoli colleghi, le vicende oggetto dell'attuale interesse dal parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ed oggi oggetto di questo intervento parlamentare sono all'attenzione del sottoscritto per diversi aspetti, che riguardano i profili connessi di natura disciplinare, organizzativa e normativa. Con particolare riferimento all'ingerenza sulle comunicazioni e attraverso esse alla conoscenza conoscenza degli spostamenti dei soggetti appartenenti ai Servizi di sicurezza e di *intelligence* dello Stato, già evidenziatisi all'esito dei primi lavori del COPASIR, deve essere intanto detto che, su iniziativa del Governo, sono in corso di discussione dinanzi alla Camera dei deputati importanti modifiche all'attuale regolamentazione della materia non solo delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti di conversazioni telefoniche, ma anche delle modalità di acquisizione dei tabulati provenienti dal traffico telefonico. Siamo certi che questo intervento legislativo contribuirà ad una più razionale disciplina dell'intero settore. Dalla vicenda oggi in esame emergono criticità e lacune del sistema normativo afferente alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e l'acquisizione dei dati provenienti dal traffico telefonico, che impongono una rapida soluzione in grado di segnare un confine preciso tra un'attività, quella di captazione di dialoghi privati e di acquisizioni di dati telefonici, che è legittimamente esercitata allorquando è funzionale ad accertamenti volti a perseguire reati ma che è certamente indebita allorquando sia ingiustificatamente diretta nei confronti di soggetti e situazioni totalmente estranei alle indagini. Il problema riguarda, evidentemente, la generalità dei cittadini in un Paese civile e democratico che garantisca, oltre che le libertà nello Stato anche le libertà dallo Stato. Tuttavia, la portata del problema si amplifica quando un'ingiustificata e generalizzata attività invasiva, avente ad oggetto la captazione di conversazioni o la ricostruzione di rapporti interpersonali attraverso i contatti telefonici, riguardi quegli stessi organi che, nelle istituzioni democratiche, sono preposti a garantire la sopravvivenza della democrazia. Le verifiche in corso presso il COPASIR sulle attività collegate ai due noti procedimenti penali pendenti presso la procura della Repubblica di Catanzaro hanno messo in luce, tra l'altro, come siano stati acquisiti i dati relativi al traffico telefonico e agli spostamenti del Direttore del SISMI, non solo senza che questi fosse indagato - tanto ha escluso il magistrato già titolare dei due procedimenti sentito dal COPASIR ma senza che vi sia alcuna traccia delle ragioni secondo le quali la ricostruzione dei dati provenienti da quelle utenze fosse utile e funzionale alle indagini in corso. È di tutta evidenza, comunque, che dati provenienti dalle utenze telefoniche del capo dei Servizi segreti militari possano contenere informazioni rilevanti per la sicurezza dello Stato. In definitiva, gli elementi acquisiti dalla vicenda di Catanzaro, alla luce della normativa vigente e salvo l'accertamento di reati la cui competenza appartiene alle procure della Repubblica cui pure quegli accertamenti sono stati trasmessi, rassegnano un quadro preoccupante sulla permeabilità degli organi di *intelligence* ed in definitiva sulla loro stessa efficienza e sul loro funzionamento. In questo senso, la relazione sui rischi per l'efficienza dei Servizi di informazione per la sicurezza, derivanti dall'acquisizione e mancata distruzione dei dati sensibili per la sicurezza della Repubblica, redatto lo scorso 12 febbraio, fotografa in maniera assolutamente efficace il quadro emergente dalle patologie proprie dell'attuale assetto normativo in materia di intercettazioni. Tale relazione del 12 febbraio, presidente Rutelli, mi sento di condividere appieno. Nel dettaglio, senza voler entrare nel merito di accertamenti in corso, appare oltremodo insostenibile che la quasi totalità degli accertamenti relativi ai traffici telefonici, e dunque ai contatti interpersonali tra soggetti estranei ai Servizi ai Servizi di *intelligence*, fossero stati demandati a consulenti privati ai quali veniva pure delegata l'architettura del complesso dell'attività investigativa. Non può non rilevarsi come affidarsi a soggetti estranei alle forze di polizia per il compimento di delicatissime attività investigative (per altro con una delega di tale generale ampiezza), coinvolgenti ampiezza), coinvolgenti la sfera di riservatezza dei cittadini, possa compromettere financo il buon andamento e l'imparzialità che devono invece sorreggere l'attività di ogni pubblica amministrazione, ivi compresa quella giudiziaria. tanto più ove tale generalizzata delega comporti inesorabilmente la creazione di delicatissimi archivi e banche dati sensibili, in ipotesi addirittura superiori a quelle in possesso alle forze di polizia, del tutto incontrollabili quando nella disponibilità di soggetti privati. Soggetti questi che, come sembra emergere dagli atti acquisiti e dalle testimonianze assunte, si muovono con fare assolutamente irrituale, sulla base di informazioni acquisite informalmente, senza regole e senza che sia possibile ricostruire i passaggi logici e procedimentali delle attività compiute. A ciò si aggiunga che, allo stesso modo, non è possibile sapere, sulla base di quanto è accertato, chi e con quali eventuali scopi ulteriori abbia preso visione dei dati acquisiti nel corso delle attività compiute. Tanto premesso, la legislazione vigente non appresta un sistema di tutele idoneo a preservare la conoscibilità dei contatti telefonici di soggetti appartenenti ai Servizi di sicurezza dello Stato, né tanto meno che impedisca un'indebita ricostruzione dei loro spostamenti. infatti l'articolo 28 della legge n. 124 del 2007, introducendo nel corpo del codice di procedura penale l'articolo 270-*bis*, ha semplicemente previsto che l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai Servizi d'informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni. Tale ipotesi, dunque, contempla una forma di tutela sui dati provenienti da soggetti appartenenti ai Servizi di sicurezza solo quando tali dati siano stati acquisiti attraverso un'intercettazione, prevedendo, al secondo comma, che terminate le intercettazioni l'autorità giudiziaria trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta dal segreto di Stato. Statuisce poi la possibilità, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di apporre il segreto di Stato e che l'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto La norma consente soltanto la tutela delle informazioni acquisite attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Nessuna protezione è apprestata, invece, ai dati provenienti dall'analisi del traffico telefonico generato da una determinata utenza e dal rilevamento della sua posizione, oggi possibile attraverso l'individuazione di tutti i ponti radio cui tali utenze si collegano. Per tali ragioni e cogliendo questa circostanza, informo il Senato che il Governo ha predisposto un intervento normativo, presto all'attenzione del Parlamento, con il quale saranno apportate significative modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale. modifiche idonee a garantire maggiori tutele ai soggetti appartenenti ai Servizi di sicurezza e, per loro, alle delicatissime funzioni svolte dagli stessi. In particolare, con la proposta di legge che intendiamo presentare al Parlamento, viene affidata esclusivamente al procuratore della Repubblica, pena la nullità del provvedimento, la richiesta di autorizzazione a disporre intercettazioni ovvero di acquisire i dati del traffico telefonico relativi ad utenze riconducibili a soggetti appartenenti al DIS, all'AISE e all'AISI. Il procuratore della Repubblica, disposto il provvedimento, deve informarne il procuratore generale e, ove non proceda personalmente, deve espressamente indicare l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'intera procedura. Sarà cura dello stesso procuratore disporre l'immediata secretazione e custodia protetta della documentazione acquisita, che dovrà essere comunque trasmessa entro un breve termine perentorio al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di verificare se taluna delle informazioni così acquisite sia coperta dal segreto di Stato. Se entro un termine di 30 giorni il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronunzia, la documentazione resterà acquisita al fascicolo processuale. Sono previste, inoltre, alcune norme ad ulteriore garanzia della riservatezza, quali i divieti di estrazione di copia della documentazione e la verifica delle modalità di secretazione e custodia anche da parte di un funzionario del DIS a ciò autorizzato dal Presidente del Consiglio: questo è l'intendimento del Governo.

sulla base di una considerazione: si fa tanto parlare della Costituzione e dei princìpi in essa contenuti, della difesa dei quali dietro ogni angolo si annunzia la presenza di un tenace sostenitore. Stiamo tentando di renderli effettivi quei principi: in particolare, anche attraverso quest'ultima proposta, stiamo rendendo concreta quella sacrosanta libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione enunciata solennemente nell'articolo 15 della Costituzione. Stiamo dando attuazione al principio secondo il quale limitazioni di libertà e segretezza possano avvenire soltanto per un atto proveniente dall'autorità giudiziaria, che sia motivato e che avvenga con le garanzie stabilite dalla legge. Attraverso la legge e i precetti in essa contenuti, indefettibili per la pacifica convivenza sociale, garantiremo una maggiore libertà e dunque una migliore democrazia. *(Applausi

che non potesse acquisire una valenza politica il fatto che la persona di cui si è parlato in quest'Aula, ossia Genchi, avesse come è stato incidentalmente ricordato anche dal senatore Quagliariello - pesantemente insinuato: è un fatto politico. Riconosco al senatore Rutelli grande trasparenza e penso che il suo lavoro comunque non sarebbe stato condizionato da nulla.

Per l'alto ruolo istituzionale che ricopre, per la sua storia politica, egli non può non cogliere la sensibilità della necessità di comunicare tempestivamente queste informazioni. Non possiamo chiudere gli occhi, non sentire e non vedere, quando si ricoprono determinati ruoli politici così delicati. Ecco perché ho chiesto la parola. Non volevo accusare nessuno, ma affrontare un discorso politico nel segno della chiarezza, che il senatore Rutelli ci ha sì fornito, ma se l'avesse fatto un attimo prima nella sua relazione, si sarebbe evitata questa parentesi - le

Grazie